L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta. Avverte

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 16 marzo 2011. Oltre al disegno di legge sulla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori - all'ordine del giorno della seduta odierna - il calendario della settimana corrente prevede la trattazione dei seguenti argomenti: eventuale seguito dei disegni di legge sulle squadre investigative comuni sovranazionali; discussione di mozioni su donne e sistema dei *media*; deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione; discussione del disegno di legge sulla parità di accesso nei consigli di amministrazione delle società quotate, ove concluso dalla Commissione; esame della Relazione della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella Regione Lazio. In relazione alla Festa nazionale di giovedì 17 marzo, la prossima settimana 1'Assemblea terrà seduta nel pomeriggio di martedì 15 e nella giornata di mercoledì 16, per 1'esame dei seguenti argomenti: disegno di legge di modifica alla legge di contabilità e finanza pubblica, già approvato dalla Camera dei deputati; mozioni sulla situazione nei Paesi del Nord Africa e Medio Oriente; ratifica della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo; altre ratifiche definite dalla Commissione affari Nella prossima Conferenza dei Capigruppo si procederà alla calendarizzazione del decreto-legge sulla Festa nazionale del 17 marzo 2011 e saranno presi in considerazione argomenti segnalati dai Gruppi di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo, del Regolamento. La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre preso atto di una lettera, inviata dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni permanenti e al Ministro per i rapporti con il Parlamento, relativa ai limiti di proponibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione di decreti-legge.

nel nostro Paese ci sono 2.995 detenute e ben 42 sono le detenute madri con figli in istituto, 43 i bambini minori di tre anni in istituto 4 le detenute in gravidanza, sempre secondo i dati del Ministero aggiornati al mese di dicembre 2010. Noi riteniamo che la dignità delle donne e i diritti inalienabili delle persone debbano essere perseguiti nella realtà, ogni giorno, attraverso la concretezza dell'agire, così come deve essere ancor più obiettivo primo e imprescindibile garantire al massimo la tutela dell'interesse e del benessere dei minori. Il provvedimento che ci accingiamo ad affrontare, il disegno di legge n. 2568 - ricordo e ribadisco - già approvato pressoché all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, fa parte degli interventi mirati a questa tutela particolare. Si tratta di una proposta accolta in maniera trasversale; prova ne è che è arrivato all'esame della Commissione giustizia del Senato con l'indirizzo positivo da parte di tutti i Capigruppo, raccogliendo pubbliche ed entusiastiche dichiarazioni di consenso anche da autorevoli rappresentanti dell'opposizione. Il provvedimento è essenziale in quanto non solo affronta nuovamente, con la finalità di potenziarli, i diritti che vanno riconosciuti alle donne madri in stato di detenzione, ma - come ricordavo - cerca di rafforzare le tutele inalienabili dovute ai figli minori di queste donne. Oggi, seppur con ritardo, anche le norme internazionali cominciano a porre in maggiore risalto l'importanza delle relazioni familiari e la cura dei figli. Nel 2008 il Parlamento europeo, anche se con ritardo, ha approvato una risoluzione che impegna gli Stati membri a tener presente nel settore carcerario le specificità femminili e a creare condizioni di vita adatte alle esigenze dei figli che vivono con il genitore detenuto. L'ordinamento italiano già prevede una serie di norme recanti misure alternative alla detenzione tradizionale per tutelare il rapporto tra detenute e figli minori e, *in primis*, la detenzione domiciliare. In più, sono già operative sul territorio nazionale una serie di strutture che favoriscono la detenzione attenuata e i servizi per l'infanzia per i bambini delle detenute madri. Ricordo, ad esempio, l'istituto a custodia attenuata per madri di Milano (il cosiddetto ICAM inaugurato nel 2006), che propone sedi esterne agli istituti penitenziari delle sezioni a custodia attenuata e la dotazione di sistemi di sicurezza non invasivi e, comunque, non riconoscibili dai bambini (niente sbarre, niente divise per la polizia penitenziaria) e strutture protette e di servizio per loro. Proprio l'8 marzo di dieci anni fa, nel 2001, venne approvata la legge n. 40 che ha posto le basi, ampliando l'operatività degli istituti del differimento dell'esecuzione della pena e della detenzione domiciliare. Questa legge ha introdotto anche due nuovi istituti, quello della detenzione domiciliare speciale e quello dell'assistenza all'esterno dei figli minori. Tuttavia, nonostante la validità del principio, che nessuno può porre in dubbio, l'applicazione di questa legge ha presentato delle lacune. In particolare, alcune di esse sono da ricondurre all'incidenza sempre maggior del fenomeno immigratorio e ai cambiamenti da esso prodotti nella società italiana, diventata sempre più multietnica. Così accade che molte mamme, soprattutto di nazionalità non italiana, non avendo un'abitazione nella quale scontare la misura alternativa degli arresti domiciliari, sono costrette a tenere i bambini con sé nelle strutture di detenzione fino al compimento, oggi, dei tre anni; circostanza che non manca di creare numerosi problemi organizzativi alle nostre strutture carcerarie, senza contare i problemi del minore e della madre. Al compimento del terzo anno dei bambini - problema non di minore conto - queste donne sono obbligate a separarsene, con ulteriore disagio dei minori, che finiscono negli istituti a essi predisposti. Al dramma delle mamme detenute si aggiunge così il trauma dei bambini che, dopo aver vissuto i primi tre anni della loro vita da carcerati, si vedono poi sottrarre improvvisamente l'affetto più caro. Il testo unificato oggi all'esame di quest'Aula, costituito da cinque articoli, nasce dal desiderio di porre un altro tassello efficace per migliorare ulteriormente la situazione attuale e l'applicazione della legge già in vigore. Esso è anche la prima risposta concreta a una volontà espressa non molto tempo fa dal Ministro guardasigilli Alfano: «Mai più bambini in carcere». Si tratta di una volontà condivisa anche da autorevoli esponenti dell'opposizione. Quella che quotidianamente vivono le mamme detenute con i loro piccoli, cari colleghi, è una condizione che questo provvedimento vuole rendere più conforme possibile ai dettami della nostra Costituzione, che all'articolo 31 ricorda che la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,

che recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». L'obiettivo è quello di favorire e facilitare la riabilitazione nella società della mamma detenuta che, è vero, ha commesso un reato, in molti casi anche grave, perché magari reiterato, salvaguardando però *in primis* il diritto ad una crescita adeguata per i bambini innocenti nei loro primi anni di vita. È proprio a proposito degli anni durante i quali i bambini hanno diritto a rimanere accanto alle loro madri che troviamo la grande novità di questo provvedimento: con l'approvazione di questo disegno di legge, infatti, i bambini potranno rimanere accanto alla mamma fino al sesto anno di età: fino, cioè, all'inizio dell'età scolare. Si tratta di una legge di buonsenso che rientra nella più ampia cornice dei diritti delle donne, ma soprattutto dei minori e che assicura ai bambini di crescere, nonostante la loro particolare e non felice condizione, in strutture adeguate, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza a cui sono sottoposte le loro madri. Una proposta di taglio così civile non deve però indurre, cari colleghi, ad una interpretazione non corretta, in quanto riteniamo fondamentale, allo stesso tempo, il principio della certezza della pena e non cerchiamo affatto di ridurre surrettiziamente l'impatto deterrente delle sanzioni per le donne che commettono reati solo perché madri. Il disegno di legge non suggerisce di togliere dal carcere le donne con figli, bensì di far scontare la pena in strutture adeguate. Quindi, dato per certo che chi commette un reato debba stare in galera o comunque in una struttura di sicurezza, che i debiti con la giustizia vadano sempre e comunque saldati, che chi è stato condannato non può farla franca (perfino una mamma), noi non vogliamo dimenticare che ciò, secondo il nostro ordinamento, debba sempre avvenire nel rispetto della dignità dei detenuti. Ancor di più, crediamo che debba esser posto in primo piano il diritto del bambino a vivere la propria infanzia come tutti gli altri coetanei più fortunati di lui. un diritto sacrosanto che non riteniamo possa essere soggetto a limitazioni. Auspichiamo pertanto che quest'Aula voglia comprenderne la profonda importanza: si potrà fare in modo che i bambini non siano costretti a vivere dietro le sbarre, condannati ma innocenti. Passo ora al dettaglio dell'illustrazione degli articoli del provvedimento. L'articolo 1 della proposta di legge all'esame di quest'Aula interviene in materia di custodia cautelare. Il comma 1 novella l'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, il cui testo attuale prevede che quando l'imputata sia donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni con essa convivente (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole) non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Nel nuovo comma si aumenta, come ho già sottolineato, da tre a sei anni l'età del bambino e, al di sotto di questa età, non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il comma 2 del medesimo articolo 1, che novella l'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale (che dispone gli arresti domiciliari), prevede la possibilità di scontare gli arresti domiciliari presso una casa famiglia protetta, se istituita. Di conseguenza, il nuovo articolo 285*-bis* del codice di procedura penale, introdotto dal comma 3,

Tuttavia, le disposizioni indicate nell'articolo 1 del provvedimento si applicano a partire dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a partire dal 1° gennaio 2014, sempre nei limiti dei posti disponibili.

attraverso l'introduzione dell'articolo 21*-ter* nell'ordinamento penitenziario, disciplina il diritto di visita al minore infermo, anche non convivente, da parte della madre detenuta o imputata (o del padre, che si trovi nelle stesse condizioni). Viene stabilito l'obbligo per il magistrato di sorveglianza in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del minore - di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all'imputata per visitare il minore malato, con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. Nei casi di assoluta urgenza il permesso è concesso dal direttore dell'istituto: questa è un'altra novità molto importante, perché accelera la possibilità per la mamma di intervenire tempestivamente in caso di gravità della malattia del proprio bambino. La disposizione stabilisce anche il diritto della detenuta o imputata (o del padre, alle condizioni indicate) di essere autorizzata dal giudice ad assistere il figlio (di età inferiore ai 10 anni, in questo caso) durante le visite specialistiche relative a gravi condizioni di salute. Il provvedimento deve essere rilasciato non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita. L'articolo 3 interviene in materia di detenzione domiciliare (articolo 47*-ter* dell'ordinamento delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni. Il comma 1, in particolare, prevede che la donna incinta, o madre di prole di età inferiore ai dieci anni con essa convivente, possa espiare la pena della reclusione non superiore a quattro anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, anche presso una casa-famiglia protetta, oltre che, come previsto dal testo vigente, nella propria abitazione o un altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza. Il comma 2, invece, interviene in materia di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni. L'attuale comma 1 dell'articolo 47-*quinquies* prevede che, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri possano espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere ai propri figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. Il nuovo comma 1-*bis*, introdotto nel provvedimento all'esame della Commissione, dispone che il terzo della pena o, almeno, i quindici anni previsti dal comma 1, possano essere espiati, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, o presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, o nella propria abitazione (o in altro luogo di privata dimora), ovvero in luogo dì cura, assistenza o accoglienza, o nelle case famiglia protette, appositamente realizzate (nel caso di impossibilità di espiazione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora). Il provvedimento comunque prevede che tali modifiche non vengano applicate nel caso di condanna per i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 4-*bis*. L'individuazione invece delle case famiglia protette è disciplinata dall'articolo 4: spetta al Ministro della giustizia, tramite decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione delle caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette e, sulla base di tali caratteristiche, l'individuazione delle strutture gestite da enti pubblici o privati idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette. Per esempio, l'ICAM di Milano nasce proprio dalla convenzione tra Stato-Regione-Provincia e Comune, tanto che poi la struttura è di proprietà della Provincia: sono 430 metri quadri sullo stesso piano, è una struttura di assoluta eccellenza. L'articolo 5, infine, individua la copertura finanziaria del provvedimento nelle risorse destinate alla realizzazione di istituti di custodia attenuata. Quindi ci si avvale della disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), che prevede una riserva di finalizzazione in favore dell'edilizia carceraria di una quota di 500 milioni di euro delle disponibilità del Fondo infrastrutture relative alla programmazione 2007-2013. alla programmazione 2007-2013. In funzione di tutto ciò e di quanto vi ho esposto stasera, confido in una rapida approvazione del disegno di legge al nostro esame nel medesimo testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche per celebrare nel migliore dei modi la giornata dell'8 marzo.

pronunciata la Camera dei deputati, con il voto favorevole del Partito Democratico. Quando si va a leggere il titolo di questa proposta di legge ("Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori") non si può che prestare un consenso, innanzitutto di carattere generale,

temporaneamente detenute ed i figli minori. Quindi abbiamo accolto favorevolmente questa proposta, anche se, quando il testo è giunto all'esame del Senato, abbiamo avuto modo di verificare che c'erano alcune lacune, alcuni nodi che rimanevano irrisolti e che, proprio per favorire i rapporti tra la madre detenuta e il bimbo, sarebbe stato opportuno intervenire con alcune modifiche. È noto che questo disegno di legge prevede delle modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Voglio ricordare in quest'Aula come, secondo il rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia realizzato dell'associazione «Antigone», nelle carceri italiane si trovino attualmente circa 2.400-2.500 donne detenute.

attualmente sono una settantina i bambini di età inferiore ai tre anni che sono in stato di detenzione assieme alle madri. Ho voluto ricordare subito questi numeri, perché quando abbiamo cominciato a discutere di questo disegno di legge all'interno della Commissione giustizia del Senato ci sono state quasi delle proteste, delle sollevazioni da parte di alcuni senatori della maggioranza, che ritenevano quasi che intervenire su questa materia volesse dire aprire le porte del carcere a chissà quali orde di detenute, a chissà quante donne detenute. I numeri

Ricordo ancora come la legge italiana preveda già delle misure alternative alla detenzione per tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori; però, come dicevo, vi sono lacune anche in relazione ai mutamenti sociali che sono nel frattempo intervenuti. Molte madri, soprattutto quelle straniere, non avendo un'abitazione dove scontare la pena sono costrette a tenere i bambini nelle strutture di detenzione fino al compimento dei tre anni; successivamente sono obbligate a separarsi dai loro figli, che finiscono negli istituti per minori.

Nella discussione in Commissione giustizia, i senatori del Partito Democratico hanno chiesto di approfondire alcuni aspetti del testo, proprio sulla base delle audizioni che sono state svolte in quella sede. È stato evidenziato, in particolare, il rischio di arrivare ad un provvedimento analogo a quello recente chiamato "svuota carceri", cioè ad un provvedimento più che altro manifesto, assolutamente vuoto, con norme destinate a rimanere inapplicate.

Si estendono le garanzie ivi previste alle straniere in relazione all'espulsione e alle altre forme di libertà personale; si modula il regime detentivo, prevedendo la detenzione domiciliare in via generale inoltre, la casa famiglia, sempre che non sussista il rischio di reiterazione del reato, ove la detenuta sia *in vinculis* per delitti di una certa gravità. Infine, la possibilità di accompagnare il figlio in ospedale non può presupporre, come presupporrebbe per il momento questo testo di disegno di legge, un imminente pericolo di vita.

era costretta ad essere sempre incinta. Ora non ci troviamo sicuramente in questa situazione, siamo in situazioni molto diverse: i numeri sono molto contenuti, ma credo proprio che il rispetto della donna, anche se detenuta, e in particolare dei bimbi imponga un approfondimento, che può essere fatto secondo l'indicazione che formuliamo come Partito Democratico nei nostri emendamenti, e credo che l'intenzione di riportare la discussione all'interno della Commissione giustizia per affrontare in maniera più adeguata temi così delicati sia

Grazia Deledda, nel romanzo «La chiesa della solitudine», scriveva: «Possibile che non si possa vivere senza far male agli innocenti?». Vorrei pormi, e porvi, questa domanda, e vorrei che oggi fossimo in grado anche di darvi una risposta approvando questo disegno di legge e consentendo che diventi legge. Infatti, anche nel più totale relativismo dei valori etici, quale quello in cui oggi viviamo, vi è sempre un'idea che scuote le coscienze di tutti, che suscita indignazione e rabbia: la condanna di un innocente alla carcerazione. Se poi questo innocente è solo un bambino, che è nato o cresce in carcere, allora l'indignazione cede il passo al richiamo alla responsabilità, ed è questo che oggi è a noi onorevoli colleghi, che il disegno di legge oggi in discussione costituisca un atto di responsabilità per un Paese civile qual è, e vuole essere, l'Italia. Siamo infatti chiamati ad approvare un testo che introduce importanti modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di rapporto tra le madri detenute ed i figli minori, ha ben ricordato la relatrice: non entro quindi nel merito specifico dei singoli articoli, ma voglio invece dare un quadro di insieme. insieme. Privare un bambino della figura materna costituisce una profonda violenza che contrasta con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e anche con l'articolo 31 della Costituzione, ma allo stesso tempo non è tollerabile che un bambino viva i primissimi anni della sua infanzia in carcere con la madre, scontando così una pena di cui non ha colpa. Questo testo è stato approvato alla Camera, lo voglio ricordare, quasi all'unanimità: 460 dei

faccia altrettanto. Per comprendere al meglio il significato e l'impatto concreto delle modifiche oggi in discussione mi pare utile dare un beve sguardo alla situazione attuale. La legge italiana prevede la sospensione obbligatoria della pena per la donna incinta e per la madre di un bambino che non abbia raggiunto un anno di età. Vi è poi la possibilità di differire l'esecuzione della pena detentiva per la madre di prole di tre anni. Ad ogni modo, si tratta solo di una sospensione, al termine della quale la donna deve e dovrà necessariamente essere in carcere con o senza il figlio, perché deve scontare la sua pena. Fino ad oggi, però, madre e figlio hanno vissuto all'interno degli istituti di pena, in appositi spazi denominati asili nido, fino al compimento del terzo anno di età. Non so quanti di voi (certamente molti),

è qualcosa che travalica qualsiasi ragionamento giuridico o posizione ideologica e rappresenta solo un'aberrazione da cancellare nel minor tempo possibile. Queste esistenze, infatti, saranno segnate per sempre. Per tutta la vita questi fanciulli dovranno fare i conti con un trauma profondo e inspiegabile poiché vivono sofferenze di cui non hanno colpa. L'analisi della realtà delle carceri offre spunti di riflessione davvero inquietanti. Secondo un rapporto predisposto da un consulente e pediatra del carcere di Como, nella maggior parte degli istituti di pena l'area nido comprende un'unica camerata (dove sono ospitate in una convivenza forzata più coppie mamma-bambino) e una cella adibita a stanza per il gioco. Nell'area nido, dunque, restano le caratteristiche strutturali del carcere: il ridotto numero di finestre dà luogo ad ambienti poco areati, scarsamente illuminati e umidi.

L'universo di questi bambini è fatto di celle, di finestre con sbarre, di lunghi corridoi con tante porte chiuse, di pareti grigie, di campanelli di allarme che suonano all'improvviso, di continuo vocio di sconosciuti. La porta blindata del carcere è il simbolo più spesso disegnato e descritto dai bambini cresciuti in carcere (anche ciò è eloquente): una porta fredda e pesante, che si apre e si chiude solo quando altri lo decidono e che emette un particolare rumore metallico, a ricordare incessantemente che quello è un luogo dove la libertà Grazie In carcere i bambini soffrono di disturbi legati al sovraffollamento, alla mancanza di spazio e sviluppano problemi di comunicazione e di relazione, oltre che inappetenza ed apatia. La neuropsichiatria infantile ci insegna che i primi tre anni di vita - ricordiamo anche i nostri - costituiscono un momento di apprendimento delle nozioni vitali i bambini imparano a camminare, a muovere le parti del corpo in modo armonico e coordinato, ad esprimere in parole i propri pensieri. Acquisiscono la percezione di sé e degli spazi e imparano a vivere nel mondo. Per questo gli specialisti del settore invitano le madri a condurre i figli in spazi aperti. Il fenomeno dei minori cresciuti in carcere non ha ampie dimensioni statistiche, ma anche se sono padri noi dobbiamo occuparci di loro. Per migliorare questo triste scenario diventa, dunque, fondamentale introdurre ipotesi alternative alla detenzione negli istituti di pena e migliorare le condizioni della detenzione nelle carceri. Altrettanto importante è estendere l'applicabilità degli arresti domiciliari. Ebbene, le odierne modifiche legislative si dirigono proprio nelle direzioni andando a integrare un processo di riforma che, come ha ricordato la relatrice, è stato avviato nel 2001. Non dobbiamo però illuderci che in questo modo riusciremo a risolvere definitivamente il problema. Stiamo compiendo un passo in avanti, ma il nostro cammino non deve fermarsi qui. L'attenzione di noi parlamentari deve essere sempre vigile sul tema! Volgendo brevemente lo sguardo al merito delle disposizioni normative, valuto positivamente l'innalzamento da tre a sei anni dell'età del bambino al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere. Qualora non sia possibile evitare la custodia cautelare, si introduce la possibilità di scontare questa misura non più in carcere, ma in un istituto a custodia attenuata per detenute madri (cosiddetto ICAM). Ricordo benissimo questa esperienza perché fu avviata quando ero assessore alle politiche sociali della Provincia di Milano. Si tratta di una struttura costituita in via sperimentale nel 2006, in esecuzione di un progetto realizzato dalla Provincia di Milano in collaborazione con il Ministero della giustizia, il Ministero dell'istruzione, la Regione Lombardia e il Comune di Milano. L'ambiente di questo tipo di istituti è accogliente ed è simile a una casa vera e propria: lo scopo è evitare che i bambini soffrano l'esperienza della carcerazione forzata. È una struttura che non ricorda in alcun modo il carcere, essendo simile ad un asilo nido in cui i bambini possono trascorrere serenamente il periodo di "carcerazione" insieme alle loro madri: vi sono camere confortevoli e luminose, ambienti personalizzati, infermeria, ludoteca, biblioteca

Grazie La frase contiene più che altro un monito: «Sapete quanto pesano le lacrime di un bambino che soffre? Più del mondo intero!». Ma noi oggi, con il provvedimento in esame (che speriamo di poter approvare e che finalmente trovi una copertura economica), possiamo ridurre questo enorme peso per i bambini e per le loro madri. Auguriamoci di poterlo fare tutti insieme! Signora

cioè il diritto al mantenimento del legame con i propri genitori da parte dei minori. Questo diritto è riconosciuto e garantito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

che, intervenendo sulla normativa del codice civile riguardante la separazione fra i coniugi, aveva affermato un principio molto importante:

Ovviamente tale problema si verifica anche quando i genitori, madre o padre, siano detenuti.

dimenticato l'argomento ed il legislatore è stato un po' disattento su questo tema. Eppure i figli di donne detenute meritano tutta la nostra attenzione.

E questo è un tema che credo non riguardi solo le istituzioni penitenziarie, ma anche la responsabilità degli enti locali, per ciò che riguarda ad esempio la politica dei servizi sociali destinati ai minori. La detenzione di un genitore o di entrambi i genitori, come tutti possiamo comprendere, interviene sicuramente come un fatto traumatico nella vita familiare, e in particolare in quella dei figli, che diventano in questo modo l'anello debole di una catena che li priva della risorsa affettiva più importante. Per questo, pur senza voler stigmatizzare la condizione dei

Molti studi hanno evidenziato, infatti, come un figlio allontanato da una madre perché in stato di detenzione sia potenzialmente più esposto poi anche ad avere problemi con la giustizia.

In questi articoli sono contenuti dei principi molto importanti, che però rischiano di rimanere delle enunciazioni di principio, qualora si decidesse, nel testo definitivo, di rimandare troppo in là l'applicazione di questa normativa. Infatti, per com'è il testo ad oggi, l'istituzione delle case famiglia e degli istituti di custodia attenuata è lasciata a provvedimenti successivi che verranno adottati,

la nostra forte preoccupazione è che collegare l'introduzione di queste misure e di questi strumenti alla realizzazione del piano carceri sia un po' come enunciare oggi un principio per lasciarlo a futura memoria. Ecco perché gli emendamenti che abbiamo presentato rispetto alla decorrenza di questo provvedimento vanno proprio nella direzione di una accelerazione

celebrare l'8 marzo pensando a poche detenute donne, condannate alla reclusione con i propri figli, mi sembra piuttosto singolare. Non entro nel merito delle celebrazioni perché il discorso è talmente vasto che in questo contesto potrebbe apparire addirittura surreale. Prendo Prendo atto che è volontà del Parlamento esprimersi proprio oggi in senso favorevole rispetto ad un atto che io giudico di mero buonismo, come si evince anche dal tono di chi è intervenuto, nei confronti di madri detenute che per la loro condotta ed il loro stato hanno condannato i figli ad essere con loro detenuti. detenuti. È vero che bisogna rispettare tutti, perché il rispetto è uno di quei valori che purtroppo si è perso, ma se si ha il diritto di essere rispettati anche in queste condizioni bisogna anche pretendere che noi donne si abbia il dovere di rispettare tutti, compresi i propri figli. È un atto che, allo stato attuale, appare più un gesto simbolico che un incisivo strumento in grado di modificare la vita delle madri carcerate che, non va dimenticato, per essere recluse debbono aver commesso delitti di particolare gravità sociale. una legge che, mi pare onesto dire, pur facendosi carico di alcune necessità di queste madri, va a salvaguardare soprattutto i diritti dei figli che, da innocenti, subiscono la sorte di un genitore che innocente non è. Conosco le strutture carcerarie - rispondo alla collega che è intervenuta prima

nella maniera più dignitosa. Mi ricordo che l'unico segno dello stare in carcere in quella specie di nido erano le grate.

(per quanto, occorre ricordare che per ogni figlio carcerato ci possono essere figli di vittime di carcerati, siano essi donne o uomini). Attualmente, in queste situazioni, molto dipende dalla sensibilità delle direzioni carcerarie. Con la presente legge si assegna a magistrati e direzioni delle carceri una discrezionalità che, a mio avviso, è eccessiva, e che, ovviamente, carica di improprie responsabilità tali soggetti. Questo congegno è uno dei benefici che potrebbe ostacolare l'approvazione dell'atto in discussione, insieme ad altre misure che appaiono

Nel contesto del principio della funzione rieducativa della pena, trovo comunque utile dare un segno di attenzione a queste donne perché riflettano sulla situazione cui hanno costretto le proprie creature, ma soprattutto penso che si stia operando per i loro figli, in modo che possano sviluppare un futuro di progresso diverso da quello esemplificato dalle loro madri. È solo in virtù dell'innocenza e per il futuro di queste creature incolpevoli che trovo in me una disponibilità a votare questo atto, con vero spirito di servizio. Signora Presidente, il disegno di legge in esame affronta un tema e un dramma che da molti anni è all'attenzione delle istituzioni e della pubblica opinione, cioè quello dei bambini che crescono fino ai tre anni dietro le sbarre del carcere: bambini detenuti, bambini costretti a condividere la pena del carcere con le proprie madri. Prima di entrare nel merito delle disposizioni contenute nella proposta, ricordo un altro 8 marzo, quello del 2001, cioè dieci anni fa, quando, per iniziativa dell'allora iniziativa dell'allora Ministro per le pari opportunità Anna Finocchiaro, con la quale mi onoro di aver collaborato all'epoca - fu approvata la legge n. 40 recante misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori. La cosiddetta legge Finocchiaro indicò i presupposti fondamentali affinché le donne con figli minori di dieci anni (e conseguentemente i bambini al di sotto dei tre anni) potevano e avrebbero dovuto evitare la pena del carcere. In base a quella proposta, tutte le detenute, indipendentemente dal reato commesso, avrebbero potuto chiedere e ottenere gli arresti domiciliari se in possesso di alcuni requisiti, come, ad esempio, l'aver scontato almeno un terzo della pena, o 15 anni, nel caso di ergastolo. La legge, che costituiva veramente un baluardo di civiltà, tuttavia è risultata largamente inapplicata: perché la gran parte delle detenute madri risultavano incriminate per reati connessi all'uso di sostanze stupefacenti e prostituzione (che sono reati tipicamente ad alto tasso di recidività), mentre proprio la recidività del reato costituisce un elemento ostativo alla praticabilità delle misure alternative alla detenzione; inoltre, perché le stesse misure alternative alla detenzione si possono applicare solo nei confronti di chi già è condannato con sentenza definitiva chi già è condannato con sentenza definitiva e dunque non già in attesa di giudizio. Considerata poi la prevalenza di madri straniere, che spesso non dispongono di un'abitazione propria dove scontare la pena domiciliare, con la legge n. quelle mamme non hanno veramente avuto altra scelta se non tenere i bambini in carcere, dunque presso di sé, fino al compimento dei tre anni. Bambini che dopo il carcere con la madre devono affrontare un trauma forte, quello della separazione, a tre anni, dalla propria madre - ancorché in carcere - e in molti casi per essere trasferiti come pacchi postali in altri istituti

spendere parole sull'aberrazione dei bambini dietro le sbarre, anche se l'intervento della collega Spadoni Urbani, da questo punto di vista, mi ha fatto un po' cambiare idea, nel senso che mi dimostra l'importanza di continuare, invece, a discuterne.

La presenza dei bambini nei luoghi di pena va veramente oltre qualunque posizione ideologica, partitica, politica, qualunque altro ragionamento di opportunità, senza per questo nulla voler togliere a tante positive iniziative sia delle amministrazioni penitenziarie (come quelle illustrate dalla collega Baio) sia delle organizzazioni di volontariato, particolarmente attive in questi campi soprattutto nelle grandi città (penso per esempio a Roma e a Rebibbia). Liberare i bambini dietro le sbarre e garantire loro il rapporto con la propria madre non soltanto è previsto da tutti i trattati internazionali sottoscritti anche dall'Italia, ma ce lo impone la nostra coscienza civile, prima di tutto ancora la natura umana di questi diritti che riguardano i minori e anche la relazione genitoriale, *in primis* quella tra madre madre e bambino o bambina in tenera età. Per tradurre in pratica il diritto di un bambino o di una bambina a stare vicino alla propria madre lontano dal carcere con l'intento di rendere effettivi i principi inapplicati della legge Finocchiaro, ho presentato in questa legislatura il disegno di legge n. 1137, che modifica la legge n. 40 del 2001 in alcuni aspetti, innanzitutto prevedendo l'istituzione di case famiglia al di fuori della struttura penitenziaria e di case famiglia protette, come *extrema* *ratio*, ad esempio nei casi di esigenza cautelare di eccezionale rilevanza da considerarsi come unica forma di restrizione applicabile quando sia coinvolto anche un minore. Stiamo parlando peraltro di casi limite, ma, in generale, per quanto riguarda le madri detenute con figli minori, di numeri limitatissimi. Quindi, le detenute potrebbero usufruire di istituti che sono già esistenti, o che potrebbero essere realizzati con modestissimi oneri a carico dello Stato - oneri irrilevanti, invece, se confrontati con i costi effettivi della detenzione in carcere - nella prospettiva di eliminare gli ostacoli che attualmente impediscono la possibilità per queste madri di espiare la pena presso il proprio domicilio. Avevo inoltre previsto di garantire al minore l'assistenza della madre di fronte all'esigenza di cure e di ospedalizzazione e, in considerazione della rilevantissima presenza di donne straniere, di intervenire fermamente sul testo unico in materia di immigrazione, ovvero sulla Bossi-Fini, che opera attraverso una sorta di automatismo del decreto di espulsione, sia che avvenga al termine dell'esecuzione della pena detentiva, sia che avvenga a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, dal non si tiene in alcun conto la circostanza di un eventuale positivo percorso di risocializzazione compiuto dalla donna detenuta. Ovviamente, si tratta di un automatismo che colpisce anche le madri con i loro bambini, bambini che sono nati in carcere o comunque che hanno vissuto in carcere la loro brevissima vita. La valutazione del «superiore interesse del fanciullo» in questo caso è giusto - a mio avviso - che si traduca nell'opportunità di rimanere in Italia.

Di questo disegno di legge, di cui sono la prima firmataria, così come di altri presentati, come quello che vede prima firmataria la senatrice Poretti, non è stato però possibile svolgere una discussione in modo approfondito qui in Senato. La Commissione giustizia e l'Aula, infatti, in pochi gironi sono state chiamate ad approvare un testo già licenziato

Innanzitutto il provvedimento in discussione, elevando l'età dei minori coinvolti da 3 a 6 anni, ottiene il paradossale effetto collaterale che saranno di più i bambini a cui non viene evitato con certezza il carcere come misura cautelare, cui saranno di più i bambini detenuti. La detenzione domiciliare speciale continuerà ad essere un beneficio esclusivo di pochissime madri con figli - come ha già dimostrato la legge n. attuale - mentre le mamme straniere, che sono la quasi totalità delle madri detenute, continueranno a rischiare l'espulsione immediata a fine pena, essendo state totalmente e completamente ignorate da questo disegno di legge in discussione. Infine, la scarsa copertura finanziaria di questa legge non consentirà di sostenere o creare case famiglia né di individuare percorsi personalizzati di reinserimento, tutto ciò che servirebbe veramente per rendere credibile l'obiettivo che la legge dice di voler perseguire. Per tutti questi motivi, e considerando che l'esiguità del numero dei minori interessati, che resta tale - come affermato dal senatore Casson - in tutte le serie statistiche storiche, permette di trovare una soluzione giusta, definitiva e certamente senza maggiori oneri rispetto a quelli della carcerazione, si consiglia di rinviare il testo in Commissione. Potremo certamente fare meglio - ne sono convinta - in Senato, e in questo modo onorare l'8 marzo delle madri in un'altra giornata meno simbolica ma più giusta e più rispettosa dei diritti dei bambini.

né con la presunzione di conoscere un argomento così delicato ed un settore così articolato. Sicuramente non può essere affrontato sul piano delle scontro ideologico o culturale, perché di mezzo non ci sono affatto le detenute madri, ma i bambini figli delle detenute madri. Già questo dovrebbe modificare di molto l'atteggiamento che questo Senato e, in genere, le forze politiche dovrebbero tenere rispetto all'argomento in questione. Diceva Fabrizio De André, in una delle sue più famose canzoni, «anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti». Io credo che nessun nessun membro della società italiana e, più in generale, globale possa considerarsi assolto del tutto di fronte a un evento criminoso. C'è certamente una differenza fra il tema della responsabilità e quello della colpa, ma sicuramente non può esserci colpa alcuna a carico di un bambino appena nato o di un bambino di pochi anni. anni. Vi racconto adesso la storia di una donna che da un mese circa, nonostante sia incinta di sette mesi e nonostante abbia un bambino di poco più di due anni, è è in carcere in una delle strutture carcerarie peggiori d'Italia, Catania Piazza Lanza. È un carcere sovraffollato, dove non ci sono asili, aree verdi dove non ci sono strutture idonee a compiere la benché minima attività di recupero e di rieducazione per gli adulti, figuriamoci per i bambini. Immaginiamo cosa possa significare imparare a camminare in uno spazio limitato e circoscritto, con una luce ridotta e con possibilità di accesso all'esterno ben determinate e anch'esse limitate e circoscritte. «Anche se voi vi credete assolti siete» (e siamo) «lo stesso coinvolti». Allora, onorevoli colleghi, credo che questa iniziativa legislativa non vada sprecata - qualche collega del Nord direbbe che piuttosto che niente è meglio piuttosto piuttosto - e che vadano cercate tutte le possibili soluzioni per far in modo che attraverso questo strumento, che è quello che ci perviene dalla Camera, si possa creare creare una condizione migliore rispetto al tema che vogliamo risolvere. Credo che rispetto alla alla condizione del bambino detenuto - questo dovrebbe essere il titolo della legge - non ci possano essere distinzioni culturali. Credo che sia necessario fare in modo che nulla vada perduto, che tutto possa essere recuperato sulla base della conoscenza dei fatti, dei luoghi e delle circostanze e delle condizioni in cui la detenzione avviene in questo momento. Non c'è dubbio, onorevoli colleghi, che pensare alla realizzazione di istituti a custodia attenuata e contemporaneamente rispettare l'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario a proposito della territorialità della pena significherebbe per il nostro Paese affrontare spese assolutamente incompatibili con le condizioni. Si verrebbe, dunque, a determinare uno scontro fra il principio che vogliamo difendere (quello d'impedire che un bambino innocente stia in carcere) e quello di evitare sprechi. Allora, probabilmente è opportuno individuare delle soluzioni alternative che rendano territorialmente eseguibile la pena e che rendano economicamente compatibile la realizzazione di queste strutture, che magari utilizzino il più possibile realtà esistenti con le opportune modifiche e gli opportuni accorgimenti. Altrimenti potremmo correre il rischio di dover concentrare le detenute madri e i detenuti figli in pochi centri d'Italia sradicandoli dal loro territorio e, dunque, facendo venire meno il diritto dei bambini non solo di stare con la propria madre, ma di stare con il proprio nucleo familiare, di vedere i nonni, gli zii, i fratelli, il padre.

atto, forse è opportuno guardare dentro il problema e magari ascoltare chi vive dentro il problema: mi riferisco agli educatori, ai dirigenti degli istituti penitenziari, agli psicologi, ai garanti dei diritti dei detenuti, che da questo punto di vista svolgono un compito importante, alle associazioni che operano all'interno delle carceri. Non si tratta, cari colleghi, di voler premiare nessuno o di voler alimentare il mondo del crimine, ma di rispettare i diritti umani: nel caso specifico, i diritti umani di un bambino

G101, che si connette perfettamente con l'argomento in questione, prevede (naturalmente, se il Governo lo riterrà opportuno) il ripristino della commissione che stava studiando alla detenzione per tutta una serie di reati. In passato, il Parlamento e il Governo avevano nominato delle commissioni che erano state presiedute dal dottor Nordio e da altri per l'individuazione di misura alternative in grado di coniugare il momento rieducativo con quello della pena. Anche nel caso delle detenute madri, un'operazione di questo genere, che vada a

di prendere atto del lavoro che tale commissione svolse a suo tempo, di utilizzarlo e di farlo diventare una proposta operativa. L'ordine del giorno G102 riguarda invece la valutazione dell'opportunità «di adottare iniziative volte a estendere la fattispecie della partecipazione al dibattimento a distanza anche nei confronti di persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario» diverso da quello in cui deve essere resa la testimonianza. Ciò perché

un sistema penitenziario come il nostro non può permettersi né sprechi né ulteriori complessità organizzative come quelle legate al trasferimento

conosco la sensibilità del Governo rispetto a tali temi: dunque, sono convinto che in qualche modo si troverà una soluzione per far sì che questo disegno di legge non sia soltanto un manifesto, ma rappresenti realmente un'opportunità per migliorare - lo ripeto - non le condizioni delle detenute, ma quelle dei bambini.

voti *bipartisan* per svuotare un testo e non per dare una soluzione pratica al fenomeno che si vorrebbe affrontare.

Questo disegno di legge, infatti, si dovrebbe occupare dei bambini, ai bambini dovrebbe essere rivolto, e non tanto alle madri. Certo, quei bambini sono in carcere perché perché hanno un'unica colpa, che davvero non dovrebbe essere loro: quella di essere figli di donne che hanno commesso un reato, che devono scontare una pena o che sono semplicemente accusate di aver commesso un reato, però, è a quei bambini che dovremmo guardare, come Parlamento e come Senato. Questa fretta di mettere all'esame oggi, nella giornata dell'8 marzo, questo disegno di legge

una legge che dovrebbe cercare di conciliare, sì, quella sicurezza della società che si deve ovviamente salvaguardare, conciliandola con i diritti dei bambini, i diritti a vivere una infanzia, non certo nelle carceri italiane.

di fallimento da parte nostra, perché chiudere nelle carceri dei bambini in presenza di numeri così esigui è davvero inspiegabile. Se quindi interveniamo di nuovo con una legge ci dovremmo occupare di quei bambini che oggi stanno nelle carceri italiane. Il problema dei bambini italiani,

(era socialista, ma deputato nel Gruppo della Rosa nel pugno). In Commissione giustizia alla Camera si riuscì ad arrivare ad un buon testo; poi, purtroppo, si interruppe la legislatura e quindi il testo non è andato avanti. Noi come radicali abbiamo subito ripresentato, sia alla Camera che al Senato, quel testo, che aveva visto - allora - l'accordo della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Si pensava di poter ripartire da lì per cercare di risolvere il problema dei bambini che oggi si trovano nelle carceri italiane: quindi, figli di nomadi, di rom e di extracomunitari. Purtroppo, invece, il testo che arriva oggi all'Aula non si occupa di quei bambini, e quindi non andrà a risolvere il problema

in ospedale e l'essere assistito, e quindi avere accanto la mamma. Ci è stato raccontato stamattina da Leda Colombini, che si occupa di questi argomenti, in occasione di una conferenza stampa

all'ospedale per continuare almeno l'allattamento. Ditemi se questa non è una situazione paradossale che in qualche modo dobbiamo andare a risolvere ad affrontare! E parliamo di numeri

soluzione simile, cioè che la detenuta è piantonata in ospedale pur di assistere il bambino che è malato e che si trova da solo? Se non serve a risolvere questi problemi pratici,

Si arriva perfino al paradosso per cui, nell'articolo 1, si dice che la custodia cautelare può essere scontata agli arresti domiciliari per madri che hanno figli da zero a sei anni. Quindi, si innalza la legge Finocchiaro, che fino ad oggi prevedeva il limite dei

carceri italiane. È una legge che entrerà in vigore nel 2014: che senso ha licenziarla così, in fretta e furia, per non cambiarla?

Signora Presidente, gli interventi che mi hanno preceduta dimostrano quanto il tema che stiamo trattando

con le cautele e con le modifiche che si riterranno necessarie. Credo sia importante che in Aula sia arrivato oggi questo disegno di legge: perché, vedete, da quanti anni se ne parla? Quando ero responsabile delle pari opportunità nel mio partito mi occupavo di questa materia. I numeri, è vero, sono sempre stati piccoli, però la tragedia cui si assisteva era lampante e sotto gli occhi di tutti. il tema si debba affrontare, perché è evidente che ci troviamo di fronte ad un bivio. La presenza di bambini innocenti in carcere infatti una pratica contraria ai diritti umani; nello stesso tempo, anche l'allontanamento del bambino dalla madre detenuta è dannoso, perché può provocare gravi traumi e danni psicologici, e soprattutto è contro natura. Questo è il tema, e questo è il problema che come legislatori siamo chiamati chiamati ad affrontare, chi con più esperienza sull'argomento per professione e chi perché lo sente come impegno sociale. La legge n. 254 del 1975 di riforma dell'ordinamento penitenziario aveva introdotto la possibilità per le detenute di tenere i figli con sé in carcere fino fino al compimento del terzo anno di età. È una norma che, nell'ottica del legislatore del tempo, rappresentava senz'altro un principio di riconoscimento del valore della maternità anche per le recluse e dell'importanza del mantenimento di uno stretto rapporto madre-bambino durante i primi anni di vita.

È stata richiamata la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia; in realtà, l'ottica, pur pregevole per allora, si rivelò poi, da un punto di vista concettuale e pratico, un'ulteriore della donna madre detenuta. È evidente che la norma non poteva assolvere ad alcuna funzione educativa, o quanto meno di effettiva tutela del rapporto

significa falsare quantomeno la relazione tra gli altri due. Se il rapporto affettivo e simbiotico con la madre, che dovrebbe rappresentare un fattore di crescita armoniosa per un bambino, si esprime infatti in un luogo chiuso, delimitato negli spazi da chiavistelli e sbarre e con aria e luce limitate, diventa il suo contrario, cioè un'oppressione reciproca. in carcere dei bambini costituiva e costituisce sempre più un grave problema, una condizione contraria ai principi di tutela dei diritti umani. È facile immaginare quanto deleteri possano essere gli effetti di una simile detenzione forzata. dimostra uno studio condotto dall'istituto penitenziario di Rebibbia, i bambini, nonostante la giovanissima età, sono perfettamente consapevoli di non vivere in una situazione di normalità. sia ammissibile che minori incolpevoli paghino per reati mai commessi e che adulti colpevoli paghino, oltre che con la detenzione, con la pena morale dell'impossibilità di essere genitori.

più volte richiamata, conosciuta come legge Finocchiaro, che prevede forme alternative alla detenzione in cella, con l'introduzione della detenzione domiciliare speciale per condannate con figli piccoli, o il rinvio obbligatorio della pena per per donne che aspettano un bambino. La legge attualmente in vigore non è applicabile a tutta la popolazione carceraria. Ci sono casi, come quelli delle donne che non hanno una fissa dimora, o di tossicodipendenti considerati recidivi, per i quali la legge stessa risulta di obiettiva, obiettiva, difficile applicazione, con la conseguenza evidente di bambini detenuti con le proprie madri. Attualmente sul territorio nazionale si contano poco più di 20 reparti, afferenti ad altrettanti penitenziari, che prevedono concretamente la possibilità per le madri detenute di scontare la pena assieme ai propri bambini. In carcere vivono 56 bambini, distribuiti in 11 istituti, dei quali il più affollato è il carcere femminile di Rebibbia, 15 casi. Il testo oggi al nostro esame trae anche ispirazione da un'osservazione attenta e continua della realtà carceraria e dalla ricca esperienza di assistenza a minori figli di madri detenute maturata sul campo da tante associazioni di volontariato. Uno dei punti salienti del provvedimento è quello della custodia cautelare. Viene innalzata da tre e sei anni l'età del bambino al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In presenza di tali esigenze si prevede la possibilità di disporre la custodia cautelare della donna che aspetta un figlio o della madre di prole di età non superiore ai sei anni

di visita al minore infermo, anche non convivente, da parte della madre detenuta imputata. Viene cioè stabilito l'obbligo per il magistrato di sorveglianza per il direttore dell'istituto di concedere il permesso alla detenuta o all'imputata di visitare il minore malato in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute e di assisterlo durante le visite specialistiche. la detenzione domiciliare e la detenzione domiciliare speciale. La novella prevede altresì che la donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente possa espiare la pena della reclusione non superiore a quattro anni, nonché la

se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri possano essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo di dimora privata, oppure in un luogo di cura per provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. Concludo, signora Presidente, evidenziando che merita una sottolineatura

va nella giusta direzione e cerca una corretta sintesi tra l'inviolabile principio della certezza dell'esecuzione della pena inflitta - che è un valore fondamentale da tutelare se si vogliono aumentare l'efficacia della giurisdizione, la tutela della sicurezza sociale e la fiducia dei cittadini nella giustizia e, dall'altra parte, l'imprescindibile salvaguardia dei minori, che non possono e non devono espiare le colpe delle proprie madri.

Rebibbia è complessivamente un buon carcere, quasi un fiore all'occhiello, ma i tagli del Governo si fanno sentire e la situazione del personale, pesantemente sotto organico, è davvero drammatica. Purtroppo, abbiamo dovuto riscontrare all'interno della struttura penitenziaria una situazione insostenibile, sia sotto il profilo del numero di detenute in relazione alla capienza, sia sotto quello della dotazione di personale, che inevitabilmente incide sulla qualità della permanenza in dette strutture da parte delle detenute. A Rebibbia, in quel momento, vi erano ben 382 detenute, a fronte di una capienza regolamentare di 274 unità, e 12 bambini di età inferiore ai tre anni, e abbiamo riscontrato una gravissima carenza di organico, attestabile intorno al 70 per cento rispetto a quanto previsto da decreto ministeriale per tale struttura. Tutto ciò compromette in modo significativo sia le attività *intramoenia* per i soggetti reclusi, e quindi il fine rieducativo che la pena detentiva dovrebbe avere, sia gli aspetti di sicurezza interna ed esterna, oltre alla possibilità di fruire dei vari servizi all'interno di detta struttura. Studi statistici evidenziano che, a livello nazionale, la situazione è analoga. Secondo il Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia, a cura dell'associazione «Antigone», sarebbero 2.385 le donne detenute, 68 delle quali madri, e 70 i bambini di età inferiore ai tre anni reclusi con loro. parlo, poi, del problema del sovraffollamento: i 206 istituti di pena italiani oggi ospitano 68.527 detenuti, a fronte di una capacità di 44.612 posti letto regolamentari Per questo il nostro ordine del giorno, che richiama espressamente l'articolo 27 della Costituzione sulla funzione rieducativa della pena, che non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative volte a colmare, con urgenza, le dotazioni organiche delle strutture penitenziarie in generale e delle case circondariali femminili in particolare, reperendo i fondi necessari per completare l'organico degli operatori penitenziari, compresi psicologi ed educatori, provvedendo altresì alla stabilizzazione delle lavoratrici precarie e delle puericultrici in particolare, anche in considerazione della loro peculiare esperienza. Chiediamo anche di disporre opportune verifiche all'interno degli istituti al fine di accertare che le condizioni strutturali e le risorse economiche, umane e strumentali disponibili siano tali da assicurare l'attuazione del diritto al lavoro in carcere, sulla base delle positive esperienze già registrate in altri paesi dell'Unione europea. Infine, chiediamo di reperire idonee risorse finanziarie per salvaguardare i livelli retributivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, nonché per l'edilizia penitenziaria, prevedendo a tal fine la realizzazione di nuove strutture ove necessario, dando priorità all'ampliamento e all'ammodernamento di quelle esistenti. Pertanto, chiediamo ai colleghi e al Governo di accogliere quest'ordine del giorno, perché si possano migliorare davvero le condizioni di vita nei penitenziari sia dei detenuti, sia degli operatori che vi operano ogni giorno con grande professionalità.

È opportuno infatti che possano vivere in luoghi più confortevoli che non il carcere, e si sono trovate delle soluzioni: case protette o istituti a custodia attenuata, arrivando fino alla

e far così presente all'Aula che, dovendo rivedere tutta la normativa, l'intero testo in esame, sarebbe opportuno concentrarci proprio sulla necessità che i figli hanno di rimanere con le proprie madri.

forse eccessiva disinvoltura, hanno revocato la potestà genitoriale ad alcune madri, madri che, talvolta, erano colpevoli solo di

possono anche dire che quell'ambiente di fortuna dove la madre tiene il figlio non è più adatto per crescere. La famiglia

che da entrambe le parti politiche hanno, da un lato sottolineato l'importanza del provvedimento in esame, dall'altra evidenziato come rispetto all'ottimo lavoro già svolto dalla Camera forse il Senato possa fare qualcosa in più. a fare riferimento alla normativa per sommi capi, a partire dall'articolo 11 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 sul cosiddetto ordinamento penitenziario che, al comma 9, consente alle detenute madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini l'amministrazione penitenziaria deve organizzare appositi asili nido secondo le modalità indicate dall'articolo 19 del regolamento di esecuzione, però non sono presenti dappertutto. L'articolo 47-*ter* della citata legge prevedeva, tra le misure alternative alla detenzione, che le detenute madri di bambini di età inferiore ai tre anni conviventi potessero espiare la pena presso la propria abitazione od in altro luogo pubblico di cura o di assistenza, entro i limiti consentiti dalla legge. L'articolo 4 della legge n.165 del 1998 ha esteso la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare alle detenute madri di bambini di età inferiore ai

già evocata in questa sede, che ha ampliato l'operatività degli istituti del rinvio obbligatorio e facoltativo della pena per madri di prole inferiore rispettivamente ad uno e tre anni, introdotto un'ipotesi speciale di detenzione domiciliare (l'articolo 47-*quinquies* dell'ordinamento penitenziario) e un'ipotesi di assistenza di figli minori all'esterno del carcere (l'articolo 21-*bis* dell'ordinamento penitenziario).

irrisolto il problema delle detenzioni delle madri di figli di età inferiore ai tre anni e quindi di quelle bambine e di quei bambini che nei fatti risultano reclusi. «Nella XIII legislatura il Parlamento ebbe la sensibilità di approvare con ampio consenso una legge finalizzata alla promozione di misure alternative alla detenzione per le madri di bambini più piccoli, ma l'esperienza e il tempo trascorso ci dicono che diversi ostacoli, anche di ordine materiale, impediscono la sua piena attuazione. Mi riferisco all'assenza di strutture di accoglienza sul territorio che facilitino la concessione delle misure alternative alla detenzione. Il Parlamento valuterà, con la fattiva collaborazione del Governo, se e in che misura sia possibile modificare le norme che impediscono la concessione di tali misure per fatti di minore allarme sociale. Ma sono, tuttavia, certo che è possibile, su questo terreno, fare qualche passo ulteriore, fino a promuovere - di concerto con gli enti locali interessati - una rete di strutture capaci di far fronte a quelle necessità di accoglienza per le madri con bambini nonché per quegli adulti che, in grave o gravissimo stato di salute, siano dichiarati "incompatibili" col carcere, ma che nel carcere restano perché non esistono strutture di accoglienza esterne». queste le argomentazioni del Ministro. E il Consiglio conclude affermando che tali argomentazioni sembrano indicare una possibilità di sviluppo che si muove nella direzione il Consiglio auspica e che potrebbe essere ulteriormente esaminata e approfondita. È appunto la situazione in cui ci troviamo attualmente perché, a fronte degli ottimi istituti che vengono introdotti con il disegno di legge al nostro esame e che toccano la custodia cautelare, il diritto di visita al minore infermo, la detenzione domiciliare, quella domiciliare speciale e l'individuazione di case famiglia protette,

e che molto bene hanno messo in rilievo le associazioni che il presidente Berselli ci ha concesso di audire, sia pure in forma molto abbreviata. Esse hanno posto problematiche che meritano approfondimento,

ma anche degli enti locali che devono, in qualche maniera, contribuire alla creazione di strutture a custodia attenuata, dei magistrati di sorveglianza e del personale dell'amministrazione penitenziaria.

Su questo siamo tutti d'accordo. Non si tratta di una sorta di amnistia occulta o di un indulto occulto, bensì di venire incontro alle sacrosante e legittime attese di questi bambini che non debbono - ripeto, non debbono - per condivisione assoluta di questo Parlamento, vivere l'esperienza del carcere. Approdato il provvedimento al Senato, in Commissione giustizia i Gruppi di maggioranza hanno ritenuto di non presentare alcun emendamento, proprio perché si riteneva che si dovessero accelerare i tempi di approvazione dello stesso, anche alla luce della doverosa calendarizzazione del provvedimento per la data odierna, che il caso vuole essere l'8 marzo, la festa della donna.

dichiarandosi ampiamente soddisfatta della circostanza che il provvedimento fosse stato calendarizzato. La stessa Presidente del Gruppo del Partito Democratico aveva da tempo avanzato richieste pressanti perché il Parlamento giungesse a questa soluzione, ampiamente condivisa.

La maggioranza ha insistito per rispettare detto termine, voluto dalla Conferenza dei Capigruppo. Abbiamo approvato entro mercoledì della scorsa settimana il provvedimento per consentirne l'approdo in Aula. Abbiamo ora appreso che ci sarebbe l'orientamento di far ritornare il provvedimento in Commissione. Al riguardo, faccio alcune osservazioni. Non pochi componenti della Commissione giustizia dei Gruppi del Popolo della Libertà e della Lega avevano sollevato perplessità sul provvedimento ma, alla luce dell'esigenza di approvarlo nei tempi previsti, avevano rinunciato a presentare emendamenti. Ora, se il provvedimento ritorna in Commissione, va da sé che deve ritornare nella sua completezza per ricominciarne l'esame in sede referente. Non faremo certamente la discussione, ma tutti i componenti della Commissione avranno la possibilità di presentare quegli emendamenti che non sono stati presentati alla luce della calendarizzazione per la data odierna del provvedimento stesso.

ma l'intero provvedimento, perché si possa riesaminarlo in quella sede. Si concederebbe a tutti i componenti della stessa la possibilità di presentare quegli emendamenti che non sono stati presentati unicamente in funzione della calendarizzazione per l'Aula del provvedimento nella data odierna.

non è stato oggetto di una trattazione approfondita in Commissione. Lo stesso collega Berselli, dando oggi conto del fatto che i senatori della maggioranza non si sono potuti esprimere a sufficienza rispetto ad una calendarizzazione già fissata per l'8 marzo, ci dà ragione in questa richiesta. È giusto infatti che, per un provvedimento che incide così pesantemente sui diritti umani dei minori, ci sia da parte di tutti tutti i componenti della Commissione giustizia, e anche di altri colleghi esterni - ho apprezzato molto, ad esempio, l'intervento del collega Fleres - la possibilità di partecipare ai lavori e dare spunti perché la legge sia resa migliore. Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, se non sono accompagnate da una attenta valutazione circa la loro applicabilità, rischiano di non essere risolutive dei problemi che oggi caratterizzano il rapporto tra i minori e le madri detenute. Quindi, resta il problema di esaminare la possibilità di finanziare la legge, che non è assolutamente presa in considerazione, e resta la necessità di dare sfogo a una serie di audizioni che non possono altro che consentire un miglioramento della legge. Voglio sottolineare che l'intento del Partito Democratico non è quello di abbattere la legge, ma quello di migliorarne il testo. Per questo, chiedo, Presidente, che si possa tornare in Commissione per due settimane

però, deve rimanere inteso che la mia richiesta, come Presidente della Commissione, è che tutto il provvedimento torni in Commissione e non soltanto gli emendamenti presentati in Aula: ciò al fine di consentire anche a quei componenti della Commissione che non avevano presentato emendamenti, o che li avevano ritirati in funzione della calendarizzazione dell'Aula,

un'approvazione unanime. Essendo convinta che si tratti di una legge che va a mettere un tassello importantissimo nel processo di riforma sul tema della tutela delle detenute delle detenute madri dei figli minori, credo che la stessa debba essere approvata il più velocemente possibile. Per lo stesso motivo, non mi sento, come il mio Presidente, di esimermi dal dare il parere positivo a che il testo ripassi in Commissione nei termini e nei modi che il presidente Berselli ha espresso. Si lavorerà cioè sull'intero provvedimento in modo da dare a tutti la possibilità di esprimersi. Spero che la dilazione serva effettivamente a produrre un testo

i legami parentali e, quindi, tra essi il più importante, quello tra madre e figlio. Tuttavia ritengo che l'approfondimento che viene richiesto oggi nella discussione generale da più parti non possa che essere utile e non possa che avere una valenza

un ulteriore periodo di due settimane per concludere l'esame del provvedimento, che sarà poi nuovamente calendarizzato in Assemblea. Il merito di questa rivisitazione sarà la Commissione giustizia a deciderlo.